sono trascorsi i tre mesi previsti dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione in ordine alle tre richieste di *referendum* promosse ai sensi degli articoli 4 e 6

non è stato raggiunto il *quorum* di un quinto dei componenti del Senato, corrispondente a sessantacinque firme, necessario per il deposito delle stesse presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione promosso nei confronti della Camera dei deputati dal tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 91 del 2016. Con ordinanza n. 91 del 23 marzo 2016, depositata in cancelleria il 22 aprile 2016 e notificata al Senato della Repubblica il 13 giugno 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso nei confronti della Camera dei deputati dal tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, con 1'ordinanza-ricorso depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 dicembre 2015. Il Consiglio di Presidenza del Senato, nella riunione del 28 giugno 2016, ha deliberato di proporre all'Assemblea del Senato della Repubblica

Noi in quest'Aula non abbiamo mai parlato di autodichia, continuiamo a nascondere la testa sotto la sabbia ma abbiamo un grandissimo problema perché l'autodichia che noi applichiamo in queste stanze comprende qualsiasi ambito sia l'amministrazione che l'autodichia legislativa. Oggi come oggi, noi dobbiamo sempre più equipararci al mondo esterno e quindi dare la possibilità ai dipendenti di potersi rivolgere al tribunale ordinario per vedersi riconosciuti i propri diritti. Noi qui abbiamo la giustizia domestica, che è composta dai dipendenti stessi e dagli organi politici, che a mio parere non potrà mai essere imparziale quanto lo sarà un giudice ordinario. Quindi il nostro voto sarà contrario.

oggi dobbiamo discutere della possibilità che il Senato, e quindi il Parlamento complessivamente, si costituisca in giudizio per difendere un principio che è basilare nell'ordinamento attuale.

condivisibile, la decisione della Corte costituzionale. Ma noi, in questa sede, operiamo in un'altra veste, siamo senatori della Repubblica e rappresentiamo l'istituzione del Senato, che comprende non soltanto i senatori in sé ma tutto Grazie, sapendo che le regole sono diverse, anche dal punto di vista della giustizia, da quelle ordinarie. Quindi siamo davanti a questo sistema. Del resto ci sono organismi che noi stessi rappresentiamo in questo contesto e ci sono colleghi che si occupano di questo. Quindi io dico che oggi dobbiamo costituirci in giudizio come ci ha proposto il Consiglio di Presidenza e ogni altra cosa si potrà valutare in prospettiva, che per la verità io neanche condividerei, ma comunque in prospettiva. Parlare oggi di cambiare le regole con un voto di questo genere è solo un atto demagogico.

Grazie,

Grazie,

da parte dei dipendenti, nei confronti appunto di Presidenti di Gruppo e altri organismi, e non vi è stata alcuna discussione né

oppure ci troviamo davanti a una situazione che vede un'applicazione molto diversificata delle norme stesse. Quindi, per tutti questi motivi, riteniamo - in questo caso tra l'altro si tratta in particolare di questioni che attengono alla tutela dei diritti dei dipendenti

Grazie, che qui sono in atto comportamenti molto diversi. Attualmente vi sono già molte cause in piedi, anche davanti alla sezione seconda lavoro di Roma, e non mi pare che il Senato abbia sentito la necessità

deliberata dal Consiglio di Presidenza. Se approvata, la Presidenza si intenderà autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, all'Avvocatura generale dello Stato. Metto ai voti la proposta

L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento RGT) nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, trasmessa dal tribunale di Campobasso». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

anzitutto bene ha fatto a sottolineare che il relatore in Giunta è stato il senatore Crimi, Grazie, un'ipotesi accusatoria relativa ad un articolo - dal titolo «L'onore dell'Italia ai parà assassinati» - nel quale sarebbe stato offeso l'onore e il prestigio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che quest'ultimo avesse ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futili, conditi da occasioni conviviali e spettacoli musicali. Per tutta una serie di ragioni che riguardano la prassi, ma anche la specificità

deliberare che le dichiarazioni rese da Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, e pertanto ricadono nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione)*.

L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Milo,

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione

mi rimetto alle sue decisioni, Presidente, ammettendo che non sono preparato, così come si dovrebbe, per sostituirlo nella relazione.

il senatore Buemi le ha comunicato che sta per arrivare, posso sospendere la seduta oppure lei sarà così cortese da fare la relazione e sostituirlo.

il senatore Milo ha parlato con un brusio dell'Aula davvero sconveniente. Quando si tratta una questione come quella ora in esame, credo che i colleghi dovrebbero ascoltare attentamente,

al vostro attento ricordo che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Milo, della quale oggi siamo chiamati ad occuparci, trova un preciso antefatto logico antefatto logico e giuridico nella precedente richiesta, da parte dello stesso ufficio giudiziario e in relazione agli stessi fatti, di autorizzazione all'acquisizione e al successivo utilizzo delle informazioni relative al posizionamento delle sue utenze cellulari, quali si desumono dai tabulati del traffico telefonico. Al relatore Buemi questo particolare, questo dato, questo antefatto logico. Che sia sfuggito al senatore Buemi, relatore, lo comprendo, ma mi stupirei molto se sfuggisse

Fatti emersi successivamente hanno provato, tuttavia, che la nostra decisione fu errata, sia pure non per scelta consapevole e volontaria dei senatori. in quell'occasione non poteva conoscere - come in effetti non la conosceva nemmeno il diretto interessato, senatore Milo - l'esistenza, nella procedura in corso nei confronti dello stesso, di gravi anomalie idonee a compromettere la stessa utilizzabilità processuale degli atti oggetto della precedente autorizzazione e di quella relazionata oggi. Il senatore Milo infatti, nell'esercizio dei suoi diritti non già di senatore si badi - ma di cittadino indagato, ha avanzato richiesta di informazioni sulla sua condizione e sui tempi e modi in cui essa fu formalizzata, sino a ricevere, non senza aver dovuto vincere ostacoli e meline

e quindi non nel modello 21 - ma la cosa non cambia - soltanto dopo che la precedente richiesta di autorizzazione - si badi, già valutata e decisa da questo consesso

soltanto dopo molti mesi, si iscrive (non già nel modello 21, ma nel SICP) il senatore Milo come indagato. Ciò vuol dire che, quando è arrivata questa richiesta il senatore Milo non risultava affatto non risultava affatto indagato, sorvola su questo dato; un dato di una rilevanza importantissima, un dato che attiene ai rapporti tra Parlamento e magistratura, tra due poteri dello Stato. Si sorvola e lo si lascia scivolare dalla penna. A giudicare dai certificati del gip di Napoli, sembrerebbe che sia stata richiesta una autorizzazione al compimento di un atto d'indagine espressamente indirizzata nei confronti di un parlamentare, senza che egli fosse stato iscritto, per quei reati per cui l'autorizzazione l'autorizzazione veniva sollecitata, nel registro di notizie di reato. Una tale mancanza, signor Presidente, non può essere banalizzata, perché essa implica, inevitabilmente, l'impossibilità di verificare e controllare il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari da parte dell'autorità giudiziaria Presidente, di una omissione gravissima, che non può non essere valutata per giudicare complessivamente le iniziative giudiziarie in corso nei confronti del senatore Milo. Sappiate, onorevoli colleghi, che il tema della verifica dei tempi di iscrizione al registro generale è incandescente e ha costretto la suprema Corte, in presenza di orientamenti contrastanti, a intervenire a sezioni unite per di cassazione, che l'iscrizione resta atto di esclusiva competenza del pubblico ministero e che non è consentito al giudice di stabilire una diversa decorrenza, fermi restando, però, gli eventuali profili di responsabilità disciplinare

nella quale i giudici di legittimità mostrano di ben comprendere la posta in gioco. Essi scrivono che: «Va solo rilevato, semmai, come, alla luce del numero delle ordinanze di rimessione (...), il problema dei possibili "arbitrii" del pubblico ministero sia stato e sia tuttora acutamente avvertito anche nella pratica quotidiana».

anche in questo caso e se sia effettivamente esigibile il rispetto delle regole anche nei confronti della magistratura e del pubblico ministero. Non sappiamo se l'omissione sia dovuta a una svista del pubblico ministero. Voglio immaginare anche un errore della sua segreteria, un incidente informatico o una certificazione errata del gip. Ma quello che non tollerabile è che il Senato possa - come in effetti ha già fatto una volta - far finta di niente, girando il capo e rifiutandosi di accertare

Da quando è iscritto? Per quali reati? Ebbene, queste domande devono essere anticipate alla fase dell'istruttoria della relazione, così da consentire ai senatori in Assemblea di non commettere altri errori, come quelli sofferti già dal senatore Milo. In questa prospettiva formulo il mio plauso, signor Presidente, ai lavori della Giunta della Camera, che pochi giorni fa ha sollecitato il rigetto di una analoga richiesta formulata dallo stesso ufficio giudiziario. Si badi: lo stesso ufficio giudiziario formula una richiesta alla Camera relativa a un deputato che non risultava iscritto nel registro degli indagati.

soltanto l'aver menzionato il nome di Bettino Craxi in un decreto di perquisizione destinato ad altri soggetti per essere sanzionato dal Consiglio superiore della magistratura ed essere poi trasferito a Trapani, dove poi ha continuato la sua attività subendo

e avendo nel massimo conto i valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, viene da dire che tra un estremo e l'altro e l'altro (un non indagato destinatario di un'autorizzazione ad acquisire i tabulati del suo traffico telefonico) c'è e ci deve essere un punto di equilibrio diverso. Deve essere in special modo evitato l'obbrobrio del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo di atti che presentino già evidenti profili di illegittimità o inutilizzabilità comuni ovvero riscontrabili a prescindere dalla qualifica di parlamentare dell'indagato, e certamente sintomatici di un'attività investigativa condotta in modo quanto meno superficiale. Sento quindi il dovere, come cittadino, come avvocato e come senatore della Repubblica di chiedere a tutti voi un convinto voto contrario all'autorizzazione richiesta all'Ufficio di Presidenza

attiene - come ha detto il senatore Milo - ai rapporti tra le istituzioni, a quel rapporto di lealtà che ci deve essere fra due poteri dello Stato. Ella, signor Presidente,

il mio intervento va nella direzione di tutelare l'organismo del quale faccio parte, il Senato della Repubblica. Mi rivolgo poi a voi, colleghi del Movimento 5 Stelle, anche voi avete il dovere di fare in modo che il nostro Senato, il nostro organismo, venga rispettato da tutti e, in particolar modo, dai componenti

fermo ma pacato invito. A voi tutti, colleghi, dico: pensateci bene, di qui a un attimo, quando voterete. State per votare un provvedimento che è strettamente collegato a uno precedente che, slealmente, ci venne richiesto e che noi, in perfetta buona fede, concedemmo

è stata formulata in un momento nel quale non era iscritto nel registro degli indagati - fatto che è stato ribadito dal senatore Falanga - credo sia interesse di tutto quanto l'emiciclo

condivido pienamente quanto detto dal senatore Quagliariello. Al di là di tutto, questa vicenda ha dell'incredibile per come si è svolta e continua a svolgersi. Io do per

autorizzazioni, già concesse, su un non indagato. Il problema è serio e, spesso, sottovalutato. Quest'Aula continua a sottovalutare argomenti seri.

Non è così. Oltretutto in questo caso vi è una ulteriore aggravante. Nulla la Camera ha dovuto pagare: nessuna truffa è stata perpetrata, perché non sono mai state consegnate Anzi, dalle stesse intercettazioni - a quanto mi risulta - è certificata la presenza del senatore Milo al centro fisioterapico: è questo il dato reale. Si tratta di un fatto incredibile, che certamente deve

ad esempio - la senatrice Bonfrisco per fatti miei, al di là di ogni regola e legge. Questo ha qualcosa di incredibile e tanti di voi, anche in questo momento, fate finta di non sentire, perché esiste un vizio e c'è paura: non si attacca chi

Poi a tutti noi spetterà decidere, in perfetta buona fede, al di là delle parti politiche, delle simpatie e antipatie. Ricordiamo che siamo, in fin dei conti, tutti esseri umani.

non si può concedere l'autorizzazione, perché è bacata alla base. Quindi, in tutta serenità e in totale autonomia, come deve avvenire in questo Senato, autonomo

Presidente, la questione illustrata nella relazione è stata posta con responsabilità e con un'attenzione particolare

tenendo conto della necessità di procedere a quegli atti istruttori doverosi in tutti i processi per arrivare ad accertare le responsabilità, Vorrei rispondere in primo luogo al collega Falanga. Non credo che il sottoscritto debba essere richiamato a posizioni di garantismo, perché tutta la sua storia parlamentare, e non solo, è improntata a principi di assoluto garantismo. Nello stesso tempo, però, devo dire con estrema franchezza che

trasmesso, a livello di conoscenza, al sottoscritto e alla Giunta - le responsabilità devono essere accertate, ma non emergono negli atti giudiziari. non è questo principalmente il nostro compito. Il nostro compito è rilevare se esistono le problematiche e le questioni che darebbero corso a un'azione di interdizione all'utilizzo delle intercettazioni.

giudiziaria procedente. Sono fermamente convinto che lo Stato ha l'obbligo di perseguire coloro che sono ritenuti i potenziali responsabili e deve accertarne la responsabilità la responsabilità attraverso il rispetto rigoroso delle regole che abbiamo scritto nella nostra Costituzione e nel nostro ordinamento subordinato. Signor Presidente, ciò non avviene

chiedo alla responsabilità dell'Assemblea una decisione definitiva sul punto. Mi pare questo un elemento critico di ordine generale, non specifico, sul quale

Presidente, com'è noto, il Movimento 5 Stelle ha da sempre avuto una posizione molto chiara in merito a quelle che sono definite le immunità parlamentari,

sede - di far sì che quelli che sono considerati e percepiti come privilegi (ma quand'anche così non dovessero considerarsi) debbano sparire, più essere riconosciuti. E questo non perché si voglia mettere il parlamentare, e la sua libertà nell'esercizio del proprio mandato elettivo, di porre in essere ogni azione politica senza ingerenze da parte di alcuno, neanche di un altro potere dello Stato, ma perché la cronaca di questo Parlamento ci racconta una storia diversa, che è quella che - a mio modo di vedere - abbiamo sentito anche oggi in Aula. Ci racconta, cioè, una storia mediante la quale ci si vuole fare scudo di quei principi per sfuggire a una responsabilità personale, che può essere anche di natura penale, che interessa qualsiasi cittadino. Avendo ascoltato alcuni interventi in discussione generale, sembra sostenersi sostanzialmente una presunta non intercettabilità in assoluto dei parlamentari. Le motivazioni che - ad esempio - il senatore Falanga ha sollevato in merito alla tempestività dell'iscrizione sul registro degli indagati - in questo caso del senatore Milo sono circostanza ben nota ai membri della Giunta, e anche ai colleghi dell'Assemblea, sol che abbiano avuto la pazienza e l'interesse di leggere la proposta rassegnata dalla Giunta stessa. stiamo parlando di cinque conversazioni telefoniche intercorse tra l'utenza del signor Alì Rashid e il senatore Milo; intercettazioni disposte nell'ambito di indagini per il reato associativo di truffa aggravata, sappiamo poi ai danni del Servizio sanitario nazionale.

il senatore Milo è stato correttamente, legittimamente, regolarmente iscritto nel registro degli indagati. Mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando. Chi vuole sostenere la la inutilizzabilità, ovvero la necessità che noi si debba denegare alla magistratura l'utilizzo di queste fonti di prova, non riesce ai miei occhi a giustificare tale è bene ricordarlo - non riuscirà a farlo neanche al di fuori di quest'Aula, ai cittadini, perché ancora una volta ci si vuole fare scudo di una misura che in astratto potrebbe anche essere comprensibile, ma che oggi non lo è, tanto più con le emergenze dello Stato,

consistenti del mondo politico con ambienti del malaffare che - anche quando non sono mafiosi come in questo caso - rappresentano ancora quel cancro della corruzione che ci sta consumando nelle nostre coscienze, nella nostra consapevolezza di essere italiani prima che a livello di aule di tribunali. La stessa relazione conferma il fatto che non vi è evidentemente alcun *fumus persecutionis*, che non è rintracciabile in alcun modo una volontà persecutoria, perché altrimenti, cari colleghi, dovremmo sostenere - anzi, è quello che voi di fatto sostenete - che chi sta commettendo reati o chi vorrà commetterne potrà tranquillamente parlare con qualsiasi parlamentare nella certezza che quelle conversazioni telefoniche non potranno mai essere utilizzate. Volete forse sostenere questo? Volete forse indurre la malavita, i corrotti, i mafiosi, chi vuole continuare a spolpare questo Paese, a dire di telefonare al senatore o al deputato, perché tanto in Giunta e nell'Aula quelle intercettazioni non saranno mai autorizzate? anche se non vi è una direzione investigativa, se cioè non si fanno indagini nei confronti del parlamentare: in questo caso stiamo parlando di intercettazioni casuali, fortuite. Volete forse sostenere questo?

nel senso che ella ha detto che la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta del senatore Buemi. Ma la correttezza della pronunzia non rileva il numero e il nome dei presenti. A quella riunione io non ero presente, essendo impegnato in altro compito istituzionale (ero in Conferenza dei Capigruppo). E, se fossi stato presente, avrei votato contro la relazione del senatore Buemi, non per i motivi di cui ai dotti interventi dei miei più illustri (in quanto essi davvero giuristi) colleghi. come ella ben sa, la giurisprudenza costituzionale in ordine alle decisioni adottate per le autorizzazioni a procedere fa riferimento a due motivazioni sostanziali o punti focali: la data di iscrizione (quindi il fatto che le intercettazioni debbano essere casuali e non causali) e il *fumus persecutionis*. In ordine al primo dei punti focali, hanno ragione il senatore Buemi e la Giunta: la direzione d'indagine è stata concretizzata in data successiva alle intercettazioni, quindi quello a cui si fa riferimento non è un dato che può essere preso in considerazione dalla Giunta, perché riguarda l'operato di un magistrato e noi non siamo chiamati a giudicare l'operato del magistrato, ma a rilevare, secondo la giurisprudenza costituzionale, se quell'operato tiene conto del rispetto di quei due punti di cui alla giurisprudenza costituzionale.

identificazioni: di tipo A, di tipo B e di tipo C. Mi si consenta la battuta forse poco rispettosa: in questo caso mi sembra proprio che sia *fumus persecutionis* di tipo D, D, come «deputati», perché l'azione di quei magistrati mi sembra più indirizzata a una persecuzione nei confronti dei deputati e dei senatori che non altro. Vengo a spiegare la forzatura della mia affermazione. Questa è la Questa è la seconda delle autorizzazioni che trattiamo nei confronti del senatore Milo. La prima era stata chiesta per poter provare, attraverso le interrogazioni rivolte

telefonica, se fosse vero che il senatore Milo si trovava in quell'ambulatorio per essere sottoposto alle cure di cui aveva chiesto il rimborso. Quest'Assemblea consentì - anche allora con il mio voto contrario - l'autorizzazione; dopo di che i magistrati si sono accorti che,

una fattura che attestava la prestazione, avrebbe potuto benissimo chiudersi l'indagine. Invece no. A questo punto, in fase successiva, visto che la sicumera con la quale la magistratura aveva indagato era stata vanificata dalla prova evidente della presenza del senatore nell'ambulatorio, è stata chiesta l'autorizzazione all'utilizzazione di cinque intercettazioni casuali. Abbiamo letto le intercettazioni, nelle quali, signor Presidente e colleghi, non è contenuto alcunché. Il senatore Milo parla con il titolare dell'azienda e dice: «Ma insomma, mi vuoi fare la fattura? Sono venuto lì,

penale: in questo caso, con discussione ampia e dottrinale sull'autodichia, dovrebbe essere la Camera dei deputati a presentare una querela per difendersi dal tentativo di

proprio per gli argomenti che in sede di replica ci ha fornito lo stesso senatore Buemi. rinviando a una questione di carattere generale, direi istituzionale, ha detto che la successione dei tempi, ovvero la cronologia della vicenda è effettivamente impropria, non meno di quanto - glielo riassumo, se me lo consente, perché lui non c'era

di un garantista collaudato come il collega e, se me lo consente, amico Buemi l'Assemblea ha avuto testimonianza diretta di come in questo caso caso la Giunta, nel suo *plenum*, avrebbe potuto aiutare il relatore a segnalare, già in sede di relazione, questa discrepanza, sulla quale poi, focoso come si addice alla sua passione e alla sua professionalità forense, l'amico Falanga ha approfondito il suo discorso. Lasciamo stare la pur efficacissima evocazione erudita del senatore Falanga della metà degli anni Ottanta, quando Carlo Palermo fu indotto in errore dalla citazione impropria di un parlamentare in un atto che non riguardava quel parlamentare.

di una sentenza della Corte costituzionale nel merito di Parlamento, intercettazioni e richieste del pubblico ministero.

originarsi. Con la stima e l'attenzione con cui ho ascoltato - ma non condiviso - i suoi argomenti, dunque al collega Buccarella: ma allora, la preoccupazione di non consentire all'opinione pubblica di ritenere che nessun parlamentare si faccia scudo di queste occasioni, consente alla magistratura procedente di farsi essa scudo di un nostro voto diverso da quello del mio Gruppo per sanare la questione, davvero sgradevole, del suo modo e, soprattutto, come ha rilevato l'amico Buemi, dei suoi tempi nel procedere? Ecco perché a me le considerazioni del senatore Buccarella non possono convincere, perché, come ha detto lui stesso con grande onestà intellettuale, il suo Gruppo - a prescindere, avrebbe detto il principe de Curtis - su questa materia vota sempre allo stesso modo. Può darsi, confesso che altrettanto a prescindere io

e quando il collega Falanga ha chiesto che si segnalasse al Consiglio superiore della magistratura

Stefano non mi crede, oltre a guardare gli atti, può chiederle al suo predecessore, senatore Pellegrino. A me la richiesta del senatore Falanga non è sembrata né impropria, né incestuosa, però mi sembra al momento prioritario un voto nello stesso senso di quello annunziato dal senatore Mario

per renderci conto che la nostra procedura, grazie alla discussione e alla relazione, è riuscita a percepire un privilegio, da parte di chi ha sbagliato modi e tempi della procedura, che un voto come quello del senatore Buccarella consentirebbe,

il suo privilegio di parlamentare, ma ci ha semplicemente resi edotti di tempi che avevano offeso i suoi diritti di cittadino. *(Applausi del

senatori Segretari di controllare se vi siano tessere abbandonate nei vari scranni

reca la discussione del documento: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti,

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta, nella seduta del 26 aprile 2016, ha respinto a maggioranza la proposta del relatore Buemi di denegare l'autorizzazione per tutte le intercettazioni. A seguito di tale reiezione, secondo prassi consolidata, si è intesa conseguentemente accolta la proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di tutte le conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi oggetto della richiesta

non senza però aver fatto sinteticamente qualche richiamo all'oggetto

nell'ambito di un procedimento penale a carico di altri soggetti per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e reati ambientali. Tra le suddette conversazioni, nove sono state intercettate su utenze in uso a Barbara Guerra e due sono state tratte da un'utenza in uso a Iris Berardi. Il gip ha riferito che, nell'ambito del procedimento n. 27883/11, nel quale non risultava indagato Silvio Berlusconi, sono state disposte intercettazioni telefoniche che hanno individuato, tra gli interlocutori più assidui dell'indagato di quel procedimento, anche tale Magnano Francesco Calogero, il quale aveva, tra le altre, numerose conversazioni telefoniche con

Il gip ha rilevato che, dal tenore delle telefonate, emergeva come il Magnano fosse impegnato in ricerche di immobili da destinare alle suddette Barbara Guerra e Iris Berardi. Il ruolo di testimoni di queste ultime e la figura del Magnano quale uomo di fiducia di Berlusconi ha imposto un approfondimento dell'oggetto delle telefonate, al fine di accertare se la contestualità delle trattative immobiliari potesse essere messa in relazione ai processi citati a carico di Silvio Berlusconi, quali fossero le finalità o se vi fossero finalità corruttive. ha sottolineato che non è stata avvertita dall'autorità giudiziaria la necessità-opportunità di avanzare una richiesta di autorizzazione preventiva alle intercettazioni dirette sulle utenze in uso al Presidente del Consiglio, giacché l'atto di indagine non era diretto ad accedere nella sfera delle comunicazioni dello stesso, ma ad entrare nella sfera di comunicazione delle intercettate e testimoni nel processo in corso a carico di Berlusconi più altri. Ad ulteriore conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, è stato rilevato che la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare Berlusconi andavano "a vuoto" e che, nell'arco di quegli otto mesi, a fronte di quasi 400 tentativi di contatto, le indagate Guerra e Berardi sono riuscite ad interloquire con l'allora parlamentare solo 29 volte. Sotto il profilo della rilevanza, il giudice per le indagini preliminari ha riferito che delle poche conversazioni ottenute dalle due donne, la maggior parte è apparsa del tutto irrilevante, esulando l'oggetto delle stesse dai fatti oggetto di indagine; altre sono apparse rilevanti a seguito della riapertura delle indagini conseguente alla trasmissione degli atti alla procura da parte del tribunale di Milano all'esito del giudizio. In particolar modo - osserva il emerso come tra l'aprile e l'agosto 2012, nel pieno svolgimento dell'istruttoria dibattimentale relativa ai processi sopra indicati - siano state intercettate alcune telefonate nel corso delle quali, alle pressanti richieste da parte delle ragazze di adempimento degli obblighi di dazione di quanto promesso, Silvio Berlusconi subordinava le dazioni concordate all'atteggiamento processuale che avrebbero tenuto le due testimoni indagate, all'epoca costituite parti civili nei suoi confronti. Il senatore Buemi, subentrato relatore in Giunta ad una prima proposta

Berardi e della Guerra, in quanto sin dall'inizio la reale direzione delle indagini sarebbe stata nel senso di captare comunicazioni telefoniche del senatore Berlusconi e

si è intesa conseguentemente accolta la proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di tutte le conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi oggetto della richiesta dell'autorità

vadano inviati al CSM per i provvedimenti disciplinari che riterrà necessario intraprendere su chi ha commesso le forzature e le illegalità che abbiamo ascoltato in quest'Aula. Barani, prendo atto che il suo intervento era sull'ordine dei lavori e non sulla discussione e le ricordo che l'articolo 19 del nostro Regolamento prescrive che «La Giunta delle elezioni è presieduta da un senatore che la Giunta elegge fra i propri membri», che «I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni». Abbiamo il cosiddetto e ormai famoso caso Caliendo che mi pare sia emblematico del rispetto di queste norme regolamentari. Pertanto, poiché l'adeguamento alle mutazioni della composizione dei vari Gruppi parlamentari

Signor Presidente, vorrei un attimo di attenzione perché stiamo procedendo in base all'articolo 68 della Costituzione e questa vicenda ha una particolarità che la rende diversa da tutte le altre. Noi qui stiamo discutendo, signor Presidente, lei me lo insegna, di intercettazioni indirette, non di intercettazioni occasionali, come abbiamo sempre fatto.

del coinvolgimento del presidente Berlusconi, ma essenzialmente della finalità di captare il presidente Berlusconi intercettando i soggetti che vengono indicati. Non lo dico io, signor Presidente, perché il presidente Stefano nel dire che il tutto nasce da un processo per truffa a carico di terze persone, forse avrebbe dovuto ricordare che - leggo il provvedimento di iscrizione fatto dal pubblico ministero Guerra Barbara viene chiamata come Cristina Battaglia, Magnano Francesco come Buongusto Alfredo, Berardi Iris come Lo Presti Rosa, ossia con nomi di fantasia grazie forse a una condivisione nel nuovo processo penale, mi auguro che questa abitudine o prassi venga eliminata), tutti incriminati - cosa che non ho mai visto e nemmeno lei, - per il seguente titolo di reato: 319-*ter*, commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al 20 marzo 2012.

Di fronte, quindi, abbiamo già elementi per dire che si fa tutto questo, secondo quanto scrive il pubblico ministero, per inderogabili ragioni di riservatezza connessa alla notorietà delle persone indagate. Vi rendete conto che le persone indagate che ho appena citato non avevano, all'epoca, alcuna notorietà e che l'unica persona nota era Silvio Berlusconi che non veniva né indicato, né citato? seguito, avviene che queste indagini e intercettazioni durano per oltre nove mesi, e nonostante i provvedimenti di proroga, come lei mi insegna, decorsi i sei mesi non sono stati mai avvisati.

perché voglio che il Senato affermi un principio, dato che a tutti noi può capitare una intercettazione indiretta. Ebbene, dopo nove mesi,

è del tutto inutilizzabile. Nel primo caso, quando riguarda le conversazioni tra gli altri, e nel non poteva dire altro, Presidente - utilizzabilità vista la carica istituzionale del Nascente e le problematiche connesse alla valutazione dell'occasionalità o no delle conversazioni telefoniche intrattenute tra le due donne.

ossia le prime due dei due gruppi riferiti alla Guerra e la prima riferita alla Berardi. Il Partito Democratico, in particolare il Capogruppo, senatore Cucca,

coscientemente valutato, dato che siamo chiamati ad applicare l'articolo 68 della Costituzione, che vi fosse consapevolezza per tutte le intercettazioni successive alle prime due,

Lei si rende conto? Solo piccola minoranza della Giunta, tre persone, era convinta della possibilità di autorizzare tutto,

decidete se autorizzarne tre, cinque, dieci o undici. Per me valgono i principi costituzionali. Abbiamo già visto un assurdo, cioè l'iscrizione nel registro degli indagati

abbiano ponderato e volutamente considerato che solo tre delle intercettazioni potevano essere utilizzate secondo una loro visione, dimenticando quello che aveva fatto il pubblico ministero e la consapevolezza iniziale di dove si voleva arrivare.

Signor Presidente, come il presidente Stefano e lei stesso avete riferito, sono stato relatore su parte di questa questione ma intervengo come membro della Giunta e voglio esprimere le più grandi perplessità. Ci sono più questioni su cui dobbiamo decidere: la prima è relativa alla nostra competenza, signor Presidente, perché all'epoca dei fatti il dottor Berlusconi era appartenente ad altra Assemblea parlamentare: era membro della Camera dei deputati. Il dottor Berlusconi, nel momento in cui viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, non è più deputato, ma non è neanche senatore di questo Parlamento e quindi credo si dovesse far riferimento alla sua condizione all'epoca dei fatti e non a una condizione successiva che oggi, per il procedimento di decadenza che è stato pronunciato negli anni scorsi, non lo rende più partecipe di questa Assemblea. Credo che sul punto dovremo essere piuttosto rigorosi. La questione dell'appartenenza precedente di membri delle due Camere, giocata, a seconda delle convenienze, su una o sull'altra Assemblea, non mi ha mai visto d'accordo alla Camera dei deputati quando ero membro di quella Giunta e non mi vede

all'attività della magistratura. Mentre nel caso precedente i colleghi hanno visto la mia difficoltà ad assumere un atteggiamento contrario, pur con un invito ad una riflessione, in questo caso sono dichiaratamente contrario a questo tipo di attività, che ha visto, in primo luogo, iscrivere il parlamentare - di cui c'è la consapevolezza - nel registro degli indagati sotto un nome di fantasia, e poi - cosa più grave - procedere per un reato inesistente, ma semplicemente con richiamo alla fattispecie di reato per accentuare la copertura per accentuare la copertura e per giustificare le intercettazioni. Ribadisco che sono convinto che lo Stato debba procedere, attraverso l'operato della magistratura, nell'azione più rigorosa per contrastare le azioni criminali di chicchessia, che non possa farlo utilizzando metodi limite rispetto al nostro ordinamento vigente, sia quello costituzionale sia quello subordinato. Questo è il punto: può essere anche il Padreterno o un povero, singolo parlamentare, come il sottoscritto, ma le leggi devono essere uguali per tutti e non ci può essere differenza.

per cui non si procedeva, sotto nomi di fantasia dei soggetti indagati con la motivazione che gli stessi soggetti, avendo una certa notorietà, potevano indurre ad attività di carattere mediatico controproducenti. Da qui, il nome di fantasia (che adesso non ricordo neanche, ma che è agli atti). Credo che il merito delle intercettazioni debba avere altro tipo di giudizio, che l'utilizzo delle stesse non possa avvenire eludendo i principi di garanzia che devono essere un baluardo

cioè 361 volte Barbara Guerra ha cercato di parlare con Berlusconi (chiamate vocali, sms e tentativi di chiamata), e soltanto in una trentina di circostanze la Guerra ha parlato effettivamente con Berlusconi. Per ciò che concerne la Berardi, solo un'utenza a questa in uso ha avuto 39 contatti telefonici con le utenze in uso a Silvio Berlusconi, e solo in due circostanze la stessa ha effettivamente parlato con quest'ultimo. che voterete per utilizzare le intercettazioni, che le quasi 22.000 telefonate intercettate sono state casualmente indirizzate a intercettare Berlusconi, che non c'entrava assolutamente niente, se non fosse che gli stessi magistrati non hanno mai negato di conoscere il legame esistente tra le intercettate e Berlusconi, perché - scrive il gip - si dispone l'iscrizione di Barbara Guerra e Iris Berardi con nomi di fantasia, al fine di evitare fughe di notizie, e lo stesso Berlusconi è iscritto col nome di Nascente. Quindi siamo in una circostanza in cui gli stessi magistrati dicono di aver violato palesemente, platealmente, tutte le regole che sono costituzionalmente scritte per garantire che un parlamentare non possa essere intercettato, se non casualmente. Se voi volete aderire alla barzelletta - per cui su circa 20.000 telefonate intercettate e su centinaia, centinaia e centinaia di telefonate indirizzate a Berlusconi per cercare di parlare con lui,

perché i colleghi sapevano benissimo (è scritto nero su bianco) che chi votava per questa utilizzazione lo faceva stracciando la Costituzione, le regole e avallando un abuso grande come una casa da parte degli inquirenti che hanno indagato e intercettato queste utenze per intercettare Berlusconi, sapendolo benissimo, quindi violando leggi e Costituzione.

anche il senatore Buccarella. anche il senatore Buccarella. Presidente, io credo che noi e i cittadini che leggeranno gli esiti di queste decisioni oggi abbiamo un diritto da tutelare, quello alla verità. Abbiamo cioè diritto di sapere semplicemente se colui che è stato il nostro Presidente del Consiglio si è reso o no responsabile di un reato particolarmente grave, che è quello di corruzione in atti giudiziari. Se quest'assunto è contestabile, allora invito i colleghi che già hanno espresso posizioni negative sulla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di queste intercettazioni telefoniche a rendere esplicito questo intendimento e possibilmente a motivarlo. Questo è l'unico interesse, cioè quello a una verità che sarà processuale, una verità nella quale l'imputato come chiunque altro - avrà tutti i diritti e i mezzi (che certamente non mancano) per potersi difendere. Quello che io immagino e che forse non tutti noi, ma la gran parte di noi in quest'Aula sapere è semplicemente questo. Ai fini di ottenere risposta a questa domanda, per la sua rilevanza culturale, politica, sociologica e probabilmente la nostra decisione non potrà che essere quella della concessione dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. con riferimento alla circostanza più volte richiamata dell'utilizzo di pseudonimi o di nomi di fantasia per le persone sotto indagine, mi dispiace contraddire il senatore Caliendo quando parlava della data del 2011 come di un periodo in cui la Berardi e l'altra indagata fossero sconosciute ai più. Se con il vostro *tablet*

delle frequentazioni dell'ex Presidente del Consiglio, tra cui anche quelle relative alle intercettazioni in parola. Evidentemente, quindi, l'utilizzo di pseudonimi o di nomi di fantasia disposto dalla magistratura inquirente era chiaramente volto, già nel 2011, alla tutela della*privacy*, quella *privacy* tante volte invocata perché presuntivamente lesa dal contenuto di intercettazioni o di altri atti d'indagine che legittimamente sono resi pubblici; quindi non è vero.

ha corrotto dei testimoni con dazioni di denaro o di beni immobili, se ha influenzato le loro testimonianze, se se ha convinto persone a revocare la costituzione di parte civile in procedimenti penali in cui le stesse erano indicate come parti offese oppure no. Solo questa è la cosa su cui i cittadini italiani hanno diritto ad avere una risposta. Oltre alle motivazioni che ho

proprio per il principio di uguaglianza e proprio perché delle prerogative parlamentari non ci si faccia scudo in maniera subdola, noi diciamo che si tratta di misure che non dovrebbero più sussistere e che purtroppo, invece, tra l'altro, vediamo confermate nella nuova struttura del "paraSenato" previsto dalle cosiddette riforme costituzionali.

determinata, rivolgendomi ai colleghi che, magari, con il voto segreto, si riterranno liberi di votare secondo coscienza, potendo anche sfuggire alle indicazioni di partito, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, al contempo invitando ad una chiamata di coscienza tutti i colleghi dell'Assemblea, affinché la domanda cui ho fatto riferimento possa avere una risposta chiara.

in base a una sentenza rispetto alla quale, nel merito, tutte le sentenze precedenti e tutte quelle successive hanno assolo gli imputati per gli stessi fatti. È un *unicum* nella giurisprudenza italiana e gli è costato l'espulsione dal Senato. Ricordo che il senatore Berlusconi è stato assolto per i fatti per i quali era finito sotto processo, con sentenza definitiva, e queste intercettazioni sono il seguito di un processo nel quale Silvio Berlusconi è stato assolto. Ricordo che, nelle centinaia di tentativi delle ragazze di chiamare Berlusconi, egli - volete dire candidamente, ingenuamente - stava parlando del procedimento civile, non di quello sulla corruzione. Rilevo che l'ex Presidente del Consiglio ancora una volta finisce nel tritacarne giudiziario e probabilmente questa vicenda finirà come le altre, con un'assoluzione. Naturalmente, però, c'è un*vulnus* che viene rivolto a un personaggio comunque importante della storia italiana, del passato e anche del futuro (e io non faccio parte del suo partito, quindi non ho alcun interesse di partito a dire questo): attraverso atteggiamenti che, nel merito, risultano chiaramente persecutori. L'opinione pubblica non è fatta solo da persone che non ragionano, ma anche da persone che vorrebbero capire i motivi per i quali si parte dalle famose cene eleganti e si finisce dentro a una una sequela di avvenimenti che per anni tengono sulla graticola un personaggio politico, arrivando perfino a violare palesemente la legge per continuare questo tipo di persecuzione. tipo di persecuzione. Va bene, è stato eliminato, il Governo è caduto, è stato emarginato, è stato espulso dal Senato; ma perché questo accanimento attraverso la violazione della legge? Questo chiedo, Presidente, ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Infatti, quando si supera il limite della ragionevolezza, è chiaro che la gente capisce che non siamo più alla ricerca di giustizia. Siamo alla ricerca di vendette che vengono giocate contro un personaggio che avrà i suoi limiti, che avrà commesso i suoi errori, ma che continua ad essere esposto a situazioni come queste che diventano irragionevoli e vanno al di là del limite, soprattutto quando prendono in giro chi deve giudicare. Il più altri. Ad ulteriore conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, è stato rilevato che la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare Berlusconi andavano

Non so se vi rendete conto delle motivazioni che spingono a continuare questo tipo di persecuzione. Voterò contro la proposta della Giunta, ricordando anche che c'era un'ampia maggioranza in Giunta che si era pronunciata per utilizzare solo cinque di queste intercettazioni e non tutte.

Grazie, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Esposito, pendente dinanzi al tribunale di Roma». La relazione della

concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

più di altre volte, di essere chiaro, non soltanto per dovere nei confronti dei colleghi, ma per interesse in questo caso legittimo, diretto e personale...

i documenti sui quali poi votiamo, nella *querelle* che intercorre tra le parti, tra l'attore e il convenuto, tra i querelanti e il querelato siano poi sottoposti al giudizio

parti di quel documento sono spiegate in modo da essere verbalizzate nel corpo centrale dei documenti attinenti alla seduta odierna e dunque sono allegati al verbale di seduta. Il senatore Stefano Esposito, secondo gli attori, quando divenne assessore della Giunta di Roma Capitale nel luglio del 2015... *(Brusio).* Senatore D'Anna, lo facciamo in due questo intervento o lo fa soltanto lei? sin dal suo insediamento egli espresse dissensi e perplessità circa la gestione dell'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma Capitale. Secondo i querelanti, a fine luglio, in occasione della sospensione di un autista della società, sanzionato per avere pubblicato su Internet un video di denuncia delle cause di mal funzionamento del servizio, Stefano Esposito dichiarò che la responsabilità dell'accaduto era tutta in capo ai vertici dell'ATAC, per i quali si ha un problema di dirigenti. Questa è la prima delle dichiarazioni alla quale i querelanti fanno riferimento. A questa se ne aggiungono tante altre, alcune rese per iscritto, altre ai microfoni di alcune radio, tra le quali Radio Roma Capitale e anche all'interno di un approfondimento di Sky Tg24.

Giunta abbiamo seguito, differentemente da altre volte, nel corso di questa legislatura, due percorsi motivatori. Uno lo abbiamo condotto alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza parlamentare. secondo me, era già di per se stesso sufficiente ed è quello di cui mi sono fatto carico di argomentare in modo

non è condiviso probabilmente nella premessa, perché nella sostanza è stato approvato il dispositivo finale. La Giunta ha cioè deliberato di proporre all'Assemblea la decisione per cui le opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito sono opinioni e, quindi, non possono essere sottoposte

dover decidere, a seguito di una dottrina che si è formata all'interno delle decisioni della Corte costituzionale, la quale a sua volta fa riferimento a precedenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, se le frasi dette dal parlamentare siano riconducibili ai criteri di libertà da parte di un parlamentare o se esse, invece,

In particolare, la Camera dei deputati, nel 2009, a conclusione di una lunga discussione sui criteri, evidenziò e si espresse nell'intenzione che fossero confrontate due esigenze: da un lato, quella di assecondare la naturale predisposizione della politica e dei suoi esponenti parlamentari a fruire

quella per cui questa prerogativa non può essere utilizzata per farsi scudo di un'attività interpersonale che si nasconda dietro l'attività parlamentare ma che invece non riguarda l'attività parlamentare propria.

esposizione formale. «L'unico limite sussistente rispetto all'applicabilità della prerogativa di insindacabilità attiene alle opinioni espresse dal parlamentare in un ambito non politico ma personale ma personale e, in quanto tale, non riconducibile in alcun modo all'esercizio delle funzioni inerenti il mandato». esempio banale: «Si pensi a titolo meramente esemplificativo al caso in cui un parlamentare offenda un vicino di casa per una lite condominiale, condominiale, evidentemente in un ambito non ricollegabile affatto all'esercizio del mandato parlamentare - e quindi debba essere - assoggettato alla disciplina penalistica comune».

l'operato deve essere riconducibile a qualcosa che abbia un significato politico; e in questo senso, visto il mandato parlamentare, deve essere riconducibile a un'attività parlamentare espressamente esplicata: quindi interventi tenuti in Aula, in Commissione, atti sindacali. Da parte nostra si rileva come tante volte questo deliberato dalla Corte Costituzionale venga considerato in un modo troppo meccanico, ragion per cui il parlamentare che in occasione di un

procinto di un periodo feriale, in Parlamento e riprendere quanto detto in Aula oppure presentare un'interrogazione.

Stefano Esposito, si ha specificatamente un'attività in tal senso

Stefano Esposito si era più volte espresso: aveva chiesto che i vertici fossero chiamati in Commissione, aveva dato ampio rilievo al suo convincimento e alla sua attività che era addirittura antecedente

comunicata alla Giunta dal presidente Matteoli e che non c'è un resoconto. È facile a questo punto eccepire che

Stefano Esposito venisse querelato per frasi dette in Consiglio di Presidenza, se questo non potesse essere testimoniato con la relativa documentazione da parte del Presidente, non si potrebbe avere la

il processo decisionale ci fanno fortemente confermare la decisione di deliberare che non si possa procedere nei confronti del senatore Stefano Esposito, perché egli ha espresso le opinioni di cui al corpo del procedimento nei suoi confronti nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

anche se la maggioranza era di Centro Sinistra e il Governo era quello di Prodi, stilammo all'unanimità un documento che costituisse il parametro da utilizzare in tutti i casi per stabilire quando le dichiarazioni fossero o non fossero insindacabili.

effettivamente di giudizi politici - perché l'attività che svolge è strettamente collegata all'attività che avrebbe svolto in Parlamento se fosse stato aperto in quella occasione.

fa diventare sindacabili le sue opinioni. Però poi abbiamo posto un paletto molto preciso: se il parlamentare, che non ha parlato in Aula, in un atto di sindacato ispettivo o in Commissione, attribuisce dall'Aula fatti determinati a un'altra persona, cioè in qualche modo la offende o la calunnia e quindi quel cittadino o un altro parlamentare si sente leso nella sua onorabilità e lo chiama in causa, quel parlamentare ne deve rispondere davanti al cittadino. Ora qui abbiamo due casi molto simili, perché sia nel caso di Stefano Esposito che nel caso di Giarrusso abbiamo due parlamentari che fuori dall'Aula hanno attribuito fatti determinati molto gravi a una terza persona, nel caso di Giarrusso addirittura a un parlamentare del PD, con accuse che hanno a che fare con l'attività mafiosa che, se

sulla base del Gruppo di appartenenza, si cambia giurisprudenza da un momento all'altro e quello che vale per un collega di un Gruppo non vale per il collega di un altro. Questo, a mio avviso, è assolutamente inammissibile, perché sarebbe veramente svilire la nostra funzione, che è precisa.

perché il parlamentare quando si esprime e quando è critico, magari con il sistema bancario o con i poteri forti, può dire cose che un cittadino fa fatica a dire perché non ha questa tutela. Il Parlamento serve per questo. E tutti sappiamo come sarebbe facile paralizzare anche un parlamentare se fosse subissato da querele e da denunce e non avesse questo scudo che gli permettesse di fare il suo dovere di parlamentare. Evidentemente alla quarta denuncia

Gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di delibera è contrario, pur comprendendo le motivazioni che hanno determinato la Giunta a maggioranza sulla proposta di riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito con riferimento alle affermazioni citate.

sedere 74 consiglieri regionali e 21 sindaci, qualora le cosiddette riforme costituzionali dovessero approdare,

nel caso del senatore Stefano Esposito, il ruolo ricoperto nel momento in cui proferiva espressioni - che, detto per inciso, sono anche probabilmente condivisibili nel merito da parte di chi parla e dal mio Gruppo - era quello di assessore al Comune di Roma. Immaginiamo cosa potrà accadere quando il consigliere regionale siederà qui, semmai questo accadrà: si toglierà il cappello di consigliere, e metterà quello di senatore o, viceversa e quando sui propri territori dirà qualcosa o voterà qualcos'altro da consigliere regionale, in virtù del suo ruolo di parlamentare potrà avvalersi anche di questo principio. È vero che già oggi la norma di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è applicata anche ai consiglieri regionali, ma la tematica analoga delle cosiddette immunità, di cui abbiamo parlato fino a poco fa, sarà invece pienamente oggetto di dibattito e di interpretazione. Pertanto, il voto del Movimento 5 Stelle sulla proposta della Giunta è contrario.

successivo, perché le garanzie costituzionali sulle opinioni espresse dai parlamentari devono essere le più ampie possibili. Stiamo vivendo un momento particolare; nel nostro Paese c'è un dibattito politico, anche a fronte di esperienze del nostro non più recente passato, ma guardando un po' all'esterno dei nostri confini, ci sono situazioni drammatiche in queste ore che ci dovrebbero portare a valutare con maggiore attenzione i principi costituzionali che sono a difesa dell'autonomia del Parlamento e a garanzia della libera espressione dei parlamentari. Richiamo semplicemente, come puro esempio, quanto accaduto nelle settimane scorse rispetto a ben 50 parlamentari dell'opposizione in Turchia (50 su 59), inquisiti per varie ragioni dall'autorità procedente, e sappiamo anche quali sono stati gli eventi successivi, che probabilmente avevano una qualche

e fare in modo che il Parlamento assuma quel ruolo che spesso invece dimentica, e cioè essere luogo di garanzia assoluta rispetto a quell'attività di critica che spesso si rende necessaria e, con altrettanta frequenza, magari è un po' sopra di tono.

che mi hanno portato ad assumere spesso atteggiamenti controcorrente, a difesa, appunto, di questo principio di garanzia, che, come ho detto già in Giunta, deve essere assoluto. Poi si può anche discutere, però credo che nel momento in cui si introducono i "se" e i "ma" i principi diventano deboli. Occorre garanzia assoluta alla libertà di espressione di coloro che svolgono la funzione parlamentare e che in qualche misura debbono mettere in campo

perché la garanzia non è a tutela dei nostri sentimenti o dei nostri affari privati. Noi, infatti, siamo qui in una funzione pubblica a garanzia di un mandato elettorale che ci è stato assegnato e che non può avere mitigazioni nella sua posizione o nella sua libertà di espressione. In questa sede, quindi, abbiamo il dovere di difendere la nostra massima libertà di espressione su qualsiasi argomento e non dobbiamo accettare neanche attività oblique - mi consentano i colleghi questa definizione magari non propria - per cui, per dare un colpo al al disturbatore, magari lo si accusa di attività che non c'entrano con quella parlamentare o con querele strumentali. Le vicende romane sono sotto gli occhi di tutti; probabilmente il senatore Esposito magari ha alzato un po' il tono, ma c'era e c'è di che alzare il tono rispetto a certe vicende che avvengono sotto i nostri

Io sono perché la tutela sia assoluta, almeno nella libertà di espressione, poi sui fatti concreti ci possono essere le flagranze di reato che dimostrano la responsabilità senza rischi di travisamento, oppure reati molto gravi che devono essere perseguiti anche se il parlamentare è in carica eccetera. Tuttavia la garanzia della libertà di espressione,

concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di

Grazie,

Presidente, proprio per le ragioni che esponevo prima, credo che la questione non riguardi solo il senatore Giarrusso; pertanto la presenza del senatore Giarrusso era una sua facoltà. Io faccio parte della Commissione antimafia, ora in missione, e sono qui in quanto relatore.

credo che dobbiamo decidere non su quanto ci dirà il senatore Giarrusso, ma sul principio che modestamente ho prima evocato: noi in questa sede non siamo proprietà privata di noi stessi; qui svolgiamo una funzione pubblica di interesse generale, a tutela degli interessi che il popolo italiano ci ha chiesto di rappresentare nel momento in cui ci ha mandato a sedere

a supporto della richiesta avanzata dal mio Capogruppo, che la richiesta del collega Giarrusso non è determinata da una mera volontà di presenza in occasione del dibattito sul provvedimento della Giunta, bensì dalla circostanza che lo stesso collega intende

delle circostanze e per esprimere la sua dichiarazione di voto. A fronte dell'impegno istituzionale, la richiesta è di posticipare alla prossima seduta possibile, al termine della missione

senatrice Puppato)*. Dico subito che sono favorevole a un rinvio in modo che Giarrusso possa difendersi. Sottolineo che è stato particolarmente sfortunato, perché anche in Giunta, dopo aver dichiarato per iscritto e messo agli atti la richiesta di insindacabilità, di fatto non si è presentato. Non so se abbia portato giustificazioni anche in quel caso, ma faccio presente che quando io, per motivi di salute, pur avendo inviato certificati medici, sono stata assente sono stata ripresa dallo stesso Giarrusso e questa è stata anche un'argomentazione che ha determinato la mia espulsione.

Ribadisco anche un altro concetto. Il senatore Giarrusso mi ha sempre rimproverata dicendo che la Giunta aveva la priorità su tutto. Quindi, non vedo perché

Abbiamo visto che nel Gruppo M5S per molto meno vengono fatti allontanamenti, spostamenti di Commissione, sospensioni ed espulsioni. In Giunta non si può e quindi prendiamo atto di questo silenzio e invito a sollecitare al più presto una nuova seduta su questo argomento in modo che il senatore Giarrusso porti le sue argomentazioni.

la relazione: «Si precisa preliminarmente che nella seduta del 6 luglio 2016 il senatore Crimi ha riferito la circostanza che il senatore Giarrusso, con una dichiarazione alla stampa, ha chiesto la non applicazione della prerogativa dell'insindacabilità».

conseguentemente, la sua presenza qui è pleonastica. Dopodiché poteva anche evitare di andare in missione con la Commissione antimafia: la sua presenza non era così eccelsa e necessaria.

L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Esposito, pendente dinanzi al tribunale di Roma». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

il senatore Mario Michele Giarrusso, a seguito di querela presentata in data 24 maggio 2015, è indagato per il delitto previsto e punito dall'articolo 595, commi 1 e 3, del codice penale, per aver offeso la reputazione dell'onorevole Maria Gaetana Greco, parlamentare in carica presso la Camera dei deputati, eletta nel Partito Democratico, comunicando con più persone, con l'aggravante di aver usato un mezzo di pubblicità. Il giudice per le indagini preliminari espone che il senatore Giarrusso ha pubblicato in data 23 maggio 2015, sul *blog* di Beppe Grillo, una dichiarazione a sua firma avente il seguente contenuto: «È inammissibile e intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in una campagna elettorale». Sempre secondo il giudice per le indagini preliminari, il senatore Giarrusso in tale circostanza avrebbe fatto riferimento alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Greco al comizio elettorale tenutosi in Piazza Garibaldi, ad Agira, il giorno 16 maggio 2015. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non poter procedere alla diretta archiviazione del procedimento, ma di dover trasmettere direttamente gli atti al Senato della Repubblica in quanto l'espressione contestata al senatore Giarrusso è stata pronunciata indubbiamente in un contesto politico, ma a suo giudizio non si ravvisa allo stato il necessario legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, tale che quest'ultima venga ad assumere finalità divulgative della prima. Lo stesso magistrato riferisce che non sembra esservi corrispondenza di significato tra l'atto esterno e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, evidenziando - in relazione a quanto chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 2015) - che non è all'uopo sufficiente un semplice collegamento tematico, una corrispondenza contenutistica parziale o un mero contesto politico. Devo ora precisare una circostanza che ci è stata comunicata nella seduta del 6 luglio 2016 dal senatore Crimi, riferita alla volontà del senatore Giarrusso, che al tempo aveva semplicemente reso una dichiarazione alla stampa proprio poche ore prima della seduta della Giunta, il quale aveva chiesto la non applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. Essendo sopravvenuto tale elemento solo in corso di seduta, la proposta conclusiva sottoposta alla Giunta è stata elaborata dal relatore tenendo conto esclusivamente delle memorie difensive consegnate agli atti dallo stesso senatore Giarrusso, con le quali veniva invece chiesta l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità attraverso la prospettazione di una serie di argomentazioni che di seguito verranno analizzate. Peraltro, lo stesso senatore Giarrusso aveva eccepito in sede processuale l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Tutto ciò premesso, si ritiene utile richiamare brevemente la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di insindacabilità, la quale individua i limiti di applicazione della prerogativa stessa, precisando che, se tali limiti venissero infranti dalle Camere in sede ermeneutica, «tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale». In particolare, la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,

tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un "legame temporale" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. Il senatore Giarrusso ha presentato due memorie difensive, la prima in data 23 giugno, la seconda in data 29 giugno. Ovviamente, signor Presidente, queste due memorie difensive, *per incidens*, si aggiungono

Soffermandosi in primo luogo sulla memoria del 29 giugno, si rileva che, alla luce della giurisprudenza della Consulta fin qui sinteticamente riportata, l'argomentazione indicata al primo punto della memoria difensiva in questione

non può trovare accoglimento, per profili attinenti ai limiti al potere istruttorio della Giunta e in particolare per l'effetto preclusivo dei predetti limiti sulla possibilità per quest'ultima quest'ultima di accertare gli elementi costitutivi del reato. Si sottolinea in proposito che, sul piano metodologico, è stato più volte affermato, in conformità con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che l'esame svolto dalla Giunta in tale ambito deve necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o no correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore interessato. La Giunta ha quindi incentrato sempre le proprie attività istruttorie in ordine alla materia in questione su tali profili, ribadendo più volte che altre valutazioni restano del tutto estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte del magistrato, come pure alla stessa configurabilità del fatto come reato.

sindacato sulla fondatezza e nemmeno sulla legittimità dell'ipotesi accusatoria. In capo alla Giunta, in altri termini, non può riconoscersi un improprio potere di condanna o di assoluzione, non potendo evidentemente la stessa utilizzare, rispetto a un caso al proprio esame, né la formula processuale che il reato non sussiste, né la formula processuale che il fatto non costituisce reato e né tantomeno la formula in base alla quale l'imputato è colpevole, essendo indiscutibile che tale potere spetti all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Peraltro, uno sconfinamento delle valutazioni della Giunta sul piano della verifica sulla sussistenza o no del reato si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle immunità previsto dalla Costituzione; queste ultime costituiscono, infatti, deroghe al principio di uguaglianza e in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato. Si osserva inoltre che, in materia di insindacabilità, le proposte della Giunta depositate in Assemblea dai diversi relatori sono risultate sempre in linea con la giurisprudenza della Consulta, anche al fine di evitare l'effetto paradossale che argomentazioni orientate *contra costitutionem* potessero vanificare in concreto la prerogativa dell'insindacabilità, aprendo la strada a conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria di fronte alla Corte costituzionale. Per tutti questi motivi, la valutazione circa la sussistenza o no del reato, oggetto del primo punto della memoria difensiva, non può trovare ingresso nell'istruttoria della Giunta e va considerata pertanto inammissibile in sede parlamentare. Nel giudizio penale di primo grado il senatore Giarrusso potrà prospettare tale tesi difensiva e sottoporre all'organo giudicante le proprie valutazioni in merito all'insussistenza - a suo avviso - del reato per indeterminatezza della persona offesa, ottenendo eventualmente, all'esito del giudizio, un'assoluzione con la formula "in quanto il fatto non costituisce reato", ovviamente se il giudice è d'accordo. La Giunta risulta invece estranea a tale ambito è importante sottolineare che tale estraneità non è motivata sulla base di profili meramente formalistici o di dettaglio, involgendo al contrario principi costituzionali fondamentali, quali innanzitutto il principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione, che costituisce un corollario del principio di eguaglianza e che può essere derogato solo in relazione ai circoscritti ambiti di operatività delle prerogative parlamentari. Un altro principio fondamentale che verrebbe leso è quello della separazione dei poteri, alla stregua del quale l'esercizio del potere valutativo in ordine alla sussistenza o no dell'insindacabilità, spettante al Senato in virtù della cosiddetta "pregiudiziale parlamentare", incontra tuttavia il limite costituzionale del corretto esercizio di tale potere, correttezza che verrebbe meno se il Senato esercitasse il suo potere al di fuori dei confini del "*quantum possit*", sconfinando in ambiti riservati al processo penale (ovviamente con tutti i conseguenti profili di contenzioso costituzionale). L'argomentazione contenuta al terzo punto della memoria difensiva, relativo alla sussistenza di una scriminante dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, risulta parimenti inammissibile in sede parlamentare. Le cause oggettive di esclusione del reato sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (articoli 50 e seguenti del codice penale). Le scriminanti, quindi, si fondano sul principio di non contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto. La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell'antigiuridicità oppure come elementi negativi del fatto, che devono quindi mancare perché il fatto costituisca reato. Ad esempio, per la configurabilità del delitto di omicidio volontario, occorre che il fatto non sia stato commesso in presenza di una situazione riconducibile alla legittima difesa, ricorrendo la quale la fattispecie dell'omicidio volontario non può appunto perfezionarsi. Rispetto a un reato di diffamazione la scriminante dell'esercizio del diritto esclude la configurabilità del reato, ossia esclude che il fatto accertato possa essere qualificato come penalmente rilevante. L'accertamento della presenza o no di una scriminante è demandato all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, l'unica alla quale nel nostro ordinamento è attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costituitivi del reato (anche di quelli "negativi", ossia l'assenza di scriminanti). Né può trarre in inganno l'attinenza della scriminante in questione alla critica politica, atteso che alla Giunta non spetta la valutazione della sussistenza di siffatto "elemento negativo" del reato, quanto semmai la valutazione che la dichiarazione espressa *extra moenia* dal parlamentare sia o no riconducibile all'esercizio di funzioni parlamentari. L'ambito teorico e metodologico delle due predette situazioni solo apparentemente risulta simile, essendo in realtà molto diverso, e in particolare nel primo caso incentrato sulla valutazione della sussistenza o no del reato. Per un principio di divisione dei poteri l'accertamento relativo al primo dei due profili richiamati spetta all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre solo il secondo spetta alla competenza del Senato. È appena il caso di precisare che la giurisprudenza ha connotato una serie di diritti di critica: si pensi, solo a titolo esemplificativo, al diritto di critica sindacale, riconosciuto ai rappresentanti sindacali dalla giurisprudenza, sia penale che lavoristica; al diritto di critica giornalistica, corollario del cosiddetto diritto di cronaca; al diritto di satira. Ma si tratta di scriminanti che, in quanto tali, devono essere fatte valere in sede processuale dal sindacalista, dal giornalista, dal politico che non sia parlamentare e infine - come nel nostro caso - dallo stesso politico parlamentare qualora non sia configurabile l'esercizio di funzioni parlamentari. A tal proposito va rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 144 del 2015, relativamente al perimetro di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, afferma testualmente: «Va, dunque, ribadita l'inaccoglibilità della tesi sostenuta dal Senato nella memoria di costituzione, secondo la quale il perimetro dell'insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse *extra moenia* andrebbe rimodulato in senso estensivo, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare, per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale». Il confine tra critica politica in senso ampio, non idonea a radicare la prerogativa dell'insindacabilità, ed esercizio della specifica funzione parlamentare emerge a chiare lettere dalla sopracitata sentenza, che peraltro riprende un orientamento costante della Consulta. della Consulta. Il secondo punto sollevato dal senatore Giarrusso nella sua memoria riguarda una sottolineatura, ossia il fatto che l'articolo sarebbe comparso sul portale del Movimento 5 Stelle, definito «portale di natura politica e rivolto alla divulgazione delle idee del Movimento».

Tale ricostruzione contrasta *in toto* con le linee interpretative enucleate dalla Consulta. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 144 del 2015, ha precisato che «il "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità (...)), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Costituzione». Nella prima lettera, inviata dal senatore Giarrusso in data 22 giugno, lo stesso allega una serie di documenti, tra i quali l'interrogazione a risposta orale del 4 febbraio 2016, relativa ai fatti verificatisi ad Agira. Su questo punto sintetizzerò la relazione,

Da questo punto di vista, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 289 del 1998, al punto 5.2, sottolinea la rilevanza dell'accertamento temporale in cui avviene l'atto parlamentare. Osserva a tal proposito la Consulta: «Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e - ciò che conta - estranea alla funzione od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un'interrogazione *ad hoc*». In altri termini, la Corte sostiene che il parlamentare potrebbe sottrarsi facilmente e indebitamente alle proprie responsabilità, presentando strumentalmente un'interrogazione *ex post*, ossia a procedimento penale iniziato. Ovviamente il relatore non intende sostenere che il senatore Giarrusso abbia avuto questo atteggiamento, ma la suddetta sentenza della Corte rende sostanzialmente sostanzialmente inutilizzabile l'atto parlamentare per via della tempistica in cui è stato presentato al fine di richiedere l'insindacabilità. Nel caso di specie, infatti, l'interrogazione è stata depositata il 4 febbraio 2016, otto mesi dopo la querela che risale al 24 maggio del 2015. Il legame temporale richiesto dalla Corte è, quindi, nel caso in questione non ravvisabile, sia per la circostanza della posteriorità dell'atto parlamentare in questione (sotto il duplice profilo della posteriorità rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, risalente al 23 maggio 2015, come pure rispetto al procedimento penale attivato a seguito della stessa), sia per il lasso temporale enorme che caratterizza tale posteriorità (otto mesi circa). Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

l'area urbana Livorno-Collesalvetti-Rosignano è da tempo colpita da recessione economica e conseguente perdita di posti di lavoro che, per dimensione e importanza delle imprese coinvolte, è da considerarsi non solo di rilevanza regionale ma anche nazionale. Le grandi imprese presenti sul territorio stanno mano a mano abbandonando il tessuto produttivo, provocando un profondo deterioramento del sistema economico. Eppure Livorno è sempre stato il principale polo industriale della Toscana, con una forte presenza di industria pesante, metalmeccanica e cantieristica. Il suo è il sesto porto commerciale italiano e il primo della Toscana e rappresenta un importante snodo commerciale di accesso ai punti europei strategici per la mobilità La profonda deindustrializzazione (amplificatasi soprattutto quando alle industrie a partecipazione statale si sono sostituite le multinazionali) ha prodotto, negli ultimi anni, un numero elevato di disoccupati, facendo precipitare sempre più verso il baratro lo strategico settore manifatturiero. Tra l'altro, la crisi imperante sembra sembra si sia trasformata in un alibi per smantellare i diritti dei lavoratori. I casi TRW e ENI sono emblematici in questo senso. Molti uomini hanno perso il loro lavoro e altrettanti rischiano di perderlo ma, per quanto il settore produttivo sia in contrazione e gli investimenti sempre minori, non significa che le due suddette multinazionali non producano profitti. E così la situazione economica livornese appare a un punto di non ritorno, mostrando come crisi economica, crisi sociale e crisi politica siano intimamente interconnesse. Oltre 300 negozi hanno chiuso dall'inizio del 2014 il tasso di disoccupazione si aggira sul 16,1 per cento. Non si può poi omettere che il territorio livornese è stato colpito anche da significativi atti di corruzione nella riconversione industriale, relativamente all'erogazione di finanziamenti. Tutto ciò ha indotto la Giunta regionale a chiedere il riconoscimento di area di crisi industriale complessa e nel gennaio del 2015 Governo, Regione Toscana e altri enti locali stipularono un accordo che riconobbe, per l'appunto, "Livorno area di crisi complessa" al pari di altre otto realtà nazionali. Richiedere il riconoscimento di area di crisi industriale complessa dovrebbe significare il poter usufruire di finanziamenti nazionali straordinari tesi ad intervenire sui fabbisogni strutturali, occupazionali, di riqualificazione delle aree interessate e soprattutto rioccupazione degli addetti in esubero. Ma nella pratica nulla di significativo è accaduto: solo cornici di indirizzo e non veri e propri interventi. Quello che i lavoratori livornesi stanno chiedendo a gran voce, senza che nulla sia stato effettivamente percepito, è che ci possa essere un utilizzo delle risorse e degli investimenti pubblici a sostegno dei bisogni e delle esigenze dei lavoratori;

vicino a Pozzolo Formigaro a difendere alcuni terreni dall'esproprio illegittimo autorizzato per la costruzione della linea TAV del terzo valico. realtà era schierata la polizia, ma fortunatamente è andato tutto bene dal punto di vista dell'ordine pubblico. occasione ci sono state delle strumentalizzazioni, come sempre, da parte della stampa e dei giornali, sull'uso della polizia. Mentre avvenivano quei fatti nei pressi di Novi Ligure, a Pozzolo Formigaro, qui in Aula veniva rimandata la calendarizzazione del reato di tortura, anche in tal caso strumentalizzando le Forze dell'ordine. veniva rimandato sulla base di accordi politici, e non certo per il merito della legge, così come viene strumentalizzato l'uso delle Forze dell'ordine, sempre per motivi politici. Questo intervento, allora, serve intanto a chiarire che siamo stanchi di queste strumentalizzazioni. Vorremmo che il Parlamento lavorasse per fare delle leggi senza strumentalizzare i fatti che avvengono all'esterno. Non lo fa questo Parlamento per gli accordi evidenti tra Alfano, Zanda e il PD, come ci sono stati in passato per le unioni civili. Solo che questa volta forse non c'era da dare la colpa a nessuno

sono meno importanti degli accordi con Alfano, Schifani, Verdini e Zanda. Forse sono meno importanti dei diritti civili. È una legge che aspettiamo da trent'anni e questo Parlamento si è comportato in maniera disgustosa - me lo lasci dire, Presidente - perché ancora una volta non abbiamo visto votare in Parlamento una legge,

la Polizia - questioni appunto marginali - per dedicarsi veramente al bene del Paese, al bene delle Forze dell'ordine, ma anche dei cittadini che sono stati vessati da funzionari di Polizia che infangano il nome della Polizia stessa e non ne fanno parte dal nostro punto di vista, e spesso sono messi

Signor Presidente, circa due ore fa ci ha lasciati Max Fanelli: guerriero di Senigallia, malato di SLA, se ne è andato dopo una lunga malattia e una progressiva paralisi che gli ha tolto la possibilità di usare il suo corpo, se non l'utilizzo di un occhio con cui comunicava. Max è morto a cinquantasei anni nella sua Senigallia. Quando, durante un'iniziativa della sua associazione benefica per i diritti dei bambini, gli sfuggì di mano il cordoncino di un palloncino d'elio, scoprì di avere la SLA. Non si lasciò mai abbattere dal degenerare della malattia e investì invece corpo e anima in una battaglia per tutti, quella battaglia diffusasi con l'*hashtag* «iostoconMax» per il raggiungimento di una buona legge sul fine vita,

ne è andato senza ricevere risposta dalla classe politica che continua a tenere in ostaggio i diritti umani delle persone. L'apertura di una discussione su una legge sul fine vita è stato forse l'unico appello del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano totalmente ignorato dalle Camere. Facciamo sentire alla vedova di Max, Monica, ai malati che chiedono di poter decidere fino alla fine della propria vita, agli oltre 60.000 firmatari della legge di iniziativa popolare sul rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità dell'eutanasia, il calore di una politica capace di affrontare i grandi temi dei diritti delle persone. Dedichiamo una buona legge a Max, a chi non c'è più, a chi è costretto ad aggiungere alle sue sofferenze l'impotenza di non essere padrone del proprio destino e di non poter decidere della propria vita. *(Applausi

Grazie,